Signor Presidente, onorevoli senatori, sono qui a riferire su due attacchi che hanno coinvolto i nostri contingenti in Libano e in Afghanistan e che hanno portato al ferimento di alcuni militari italiani. Il primo si è verificato nel pomeriggio del 27 maggio, quando un mezzo italiano del contingente UNIFIL, mentre percorreva il tratto stradale tra Beirut e Shama, all'ingresso dell'abitato di Sidone, veniva investito dall'esplosione di un ordigno, che provocava il ferimento dei sei militari italiani trasportati a bordo. Il secondo attacco, invece, è avvenuto nella mattinata del 30 maggio, contro la base del PRT, cioè l'organismo di ricostruzione provinciale di con ordigni esplosivi e fuoco diretto che hanno causato il ferimento di cinque militari italiani. Signor Presidente, onorevoli senatori, fatta questa premessa, passo a descrivere i fatti secondo la ricostruzione effettuata dalle competenti organizzazioni tecnico-operative e sulla base delle notizie ad oggi disponibili. Il 27 maggio, alle ore 16,55 locali (mancavano cinque minuti alle ore 16 in Italia), un convoglio logistico del contingente italiano composto da quattro mezzi, un gippone VM-90, un autoscarrabile APS-95, un autosoccorso ISOLI e un altro gippone VM-90, durante un trasferimento veniva coinvolto nell'esplosione di un ordigno, verosimilmente comandato a distanza, che investiva l'ultimo veicolo della colonna. Il movimento era finalizzato a far rientrare i quattro mezzi, provenienti da Beirut, nella nostra sede, dopo che erano stati portati nelle autofficine di Beirut per la normale manutenzione. Al momento dell'evento, il convoglio si trovava al di fuori dell'area di operazione e di responsabilità di UNIFIL, che si estende a Sud del fiume Litani fino alla cosiddetta *Blue Line*, che segna la linea di confine con Israele. Tutti i movimenti al di fuori dell'area di operazione sono preventivamente autorizzati dal comando di UNIFIL, che ne stabilisce le norme di sicurezza e ne valuta, di volta in volta, la fattibilità. Nel caso in esame, questo è avvenuto: il movimento era stato regolarmente autorizzato nei modi e nei tempi in cui poi si è effettivamente svolto. Con riguardo alle misure di sicurezza, i VM-90 di testa e di coda erano equipaggiati con disturbatori elettronici, il cui uso è stato disposto dalle Forze armate italiane in aggiunta alle misure di sicurezza standard previste dal Il nostro personale si è attenuto alle norme di sicurezza in vigore che, nella specifica situazione di stato di allerta (codice giallo, ovvero livello medio-basso), prevedevano di portare al seguito, oltre all'armamento, l'equipaggiamento individuale di protezione, ossia il giubbetto antiproiettile e l'elmetto. disposal*) della *Joint task force Lebanon*, che ha condotto una prima analisi, ha appurato che l'ordigno, collocato al margine sinistro della carreggiata, è stato occultato posizionandolo nello spazio lasciato tra le barriere di protezione del tipo New Jersey che separano i due sensi di marcia. Al momento sono in corso le verifiche e gli accertamenti per determinare la tipologia e le caratteristiche tecniche dell'ordigno. L'esplosione ha provocato il ferimento di tutti i sei militari che occupavano il mezzo, dei quali non sono stati resi noti i nomi per evidenti ragioni di tutela della *privacy* e della sicurezza. In particolare, comunque, i feriti sono un sergente capo macchina, che ha riportato escoriazioni multiple del volto con ematoma periorbitario all'occhio sinistro; caporal maggiore, che ha riportato escoriazioni multiple del volto con ematoma periorbitario sinistro e del meato acustico omolaterale; un caporal maggiore capo, che ha riportato escoriazioni multiple del volto, ipoacusia auricolare destra e un trauma distorsivo contusivo un caporal maggiore che ha subìto una ferita lacero-contusa all'emitorace sinistro ed escoriazioni multiple del volto; un caporal maggiore capo che ha subìto escoriazioni multiple del volto con ematoma perioculare, lacerazione della vena giugulare trattata chirurgicamente, lacerazione dell'arteria tiroidea superiore trattata chirurgicamente; un caporal maggiore conduttore che ha riportato lesioni complesse all'emivolto sinistro con possibile compromissione delle ossa della base cranica, l'esplosione del globo oculare sinistro,

il più rapidamente possibile e quelli dei due feriti più gravi sono stati trasportati a Sidone, accompagnati da un colonnello medico dell'ospedale militare del Celio. Nei giorni successivi, non appena possibile, si è provveduto al rientro di tutti i militari coinvolti in Italia; attualmente sono ricoverati presso il

la vitale via di comunicazione e rifornimento che collega questa con la città di Beirut, ovvero che consente l'accesso ai principali porti ed aeroporti del Libano. In tal senso, il fatto che un considerevole numero di convogli UNIFIL percorrano la suddetta via regolarmente, con un notevole numero di automezzi civili, fa capire il contesto in cui quell'evento si è verificato.

solo in una precedente occasione si è verificato un simile evento - l'8 gennaio del 2008 - con il ferimento, quella volta, per fortuna, in modo leggero di 2 militari irlandesi. Ne è stato vittima, con modalità analoghe, un veicolo fuoristrada con insegne ONU a circa soli 500 metri di distanza dal luogo nel quale sono stati attaccati i nostri militari. In questo momento è prematura qualsiasi ipotesi o speculazione su motivi specifici, finalità e matrici dell'atto. E' bene per questo attendere che siano disponibili le risultanze delle inchieste in atto di UNIFIL, delle autorità libanesi e di quelle nazionali. Oggi in prima istanza, come peraltro formalmente dichiarato dal portavoce di UNIFIL, si può escludere che si sia trattato di un attacco deliberato contro il contingente italiano. E' piuttosto probabile che si sia trattato di un attacco condotto contro UNIFIL in quanto forza di stabilizzazione e di pace presente in un contesto di crisi e, pertanto, obiettivo da sempre di terroristi che hanno la volontà di destabilizzare la situazione. Va aggiunto come i veicoli di UNIFIL non siano contraddistinti con segni delle singole nazionalità, ma accomunati dal colore bianco e dalle insegne dell'ONU. Per un'analisi a carattere generale deve essere sottolineata l'instabilità dell'area mediorientale, in particolare la perdurante, complessa e fragile situazione libanese. Basti citare al riguardo questi fattori. In primo luogo, vi è l'irrisolta questione palestinese e la presenza di numerosi campi profughi in Libano, al cui interno non possono operare le forze di sicurezza libanesi. In particolare, nelle vicinanze della città di Sidone, si trova un importante campo profughi palestinese, denominato Ain El Helwi, che rappresenta una potenziale fonte di rischio nell'area per la presenza segnalata di cellule terroristiche. In secondo luogo, la situazione di crisi che interessa la Siria, Stato da sempre collegato da correlazioni di causa ed effetto con il Libano, sicuramente può essere uno dei fattori da prendere in considerazione. L'instabilità politica ed amministrativa del Libano,

vi è la persistenza di quelle stesse condizioni che hanno portato alla creazione di UNIFIL quale forza per il mantenimento della cessazione delle ostilità e per sostenere il cessate il fuoco, evento quest'ultimo che finora non è stato mai possibile conseguire in maniera integrale e che rappresenta, di per se stesso la ragione principale dell'instabilità nell'area. Concludo con il primo incidente, sottolineando il ruolo svolto da UNIFIL in generale e dal nostro contingente per il mantenimento della stabilità e della pace nell'area, come ripetutamente ribadito sia dai libanesi che dagli israeliani, oltre che dalla comunità internazionale tutta. Ciò detto, il Governo - a prescindere quindi da questo evento, e a prescindere dal ruolo di UNIFIL - sta valutando da tempo l'opportunità di una razionalizzazione del nostro contingente in Libano che, oggi, è ancora il più numeroso. Non si tratta assolutamente della volontà di ritirare il contingente. Noi restiamo fedeli al principio *"together in - together out":* insieme con le organizzazioni internazionali siamo entrati nella missione e solo in accordo con le organizzazioni internazionali ne potremo uscire. Si tratta invece di razionalizzare la nostra presenza perché, avendo ceduto ormai da tempo il comando, prima affidato al generale Graziano, al contingente spagnolo, riteniamo che essa in termini quantitativi debba subire una modifica. Abbiamo già attuato riduzioni in termini di uomini (250 circa in meno), ma riteniamo che ancora oggi la presenza di quasi 1.700 uomini sia eccessiva rispetto all'equilibrio delle altre forze nazionali che fanno parte del contingente. Da tempo si è dichiarata la nostra volontà quanto meno di arrivare ad un livello uguale a quello spagnolo, che esprime il comandante, che è di circa 1.000 uomini. L'entità del nostro contingente potrebbe quindi attestarsi su quella cifra. Ovviamente sarà necessario adottare opportune iniziative in ambito ONU per individuare opzioni compensative, ad esempio ricercando nuovi Paesi che mettano a disposizione aliquote di militari per mantenere gli attuali livelli di uomini in UNIFIL. quindi ribadire il presupposto più volte espresso che l'Italia continuerà a contribuire in modo significativo alla missione di pace e sicurezza in Libano fintanto che nell'ambito delle organizzazioni internazionali non verranno prese nuove e diverse decisioni. Passo ora a descrivere l'attacco alla sede del PRT di Herat in Afghanistan, su base del 132° reggimento artiglieria Ariete. Sulla base delle informazioni in nostro possesso in questo momento, e che dovranno essere confermate dall'inchiesta in atto, l'attacco si è verificato il 30 maggio alle ore 11,15, ovvero 8,45 italiane, ed era stato preceduto dall'esplosione di una moto - una motobomba per l'esattezza - presso l'ospedale civile di Herat, probabilmente con scopi diversivi. Dopo pochi minuti, un camioncino di colore bianco Mazda, tipo Titan, carico di sacchi di cemento e sabbia, si è presentato ad un posto di controllo che regola i movimenti sulla strada lungo il lato Sud di Camp Vianini, sede del PRT, verosimilmente accompagnato da due motociclisti che avrebbero distratto il personale di guardia dell'agenzia di sicurezza afgana *Serv Cor Security* posto a presidio del *check point*, consentendo all'automezzo di riprendere il movimento lungo la serpentina di ingresso per tentare di sfondare il portone principale del *compound* dove ha sede il PRT. Il veicolo, penetrato oltre il posto di controllo, ha superato l'ingresso sud dell'insediamento militare ed è andato ad esplodere lungo il muro di recinzione a pochi metri di distanza. Chi ha avuto occasione di visitare Herat sa che le vie intorno sono chiuse e per accedere a quelle vie, che possono anche anche condurre ad altri punti e non solo alla sede del PRT, c'è una prima porta e una prima fase di controllo. L'azione quindi non è riuscita per il complesso di misure esistenti e il camioncino non è riuscito a centrare la porta di ingresso andando a sbattere, esplodendo, contro il muro esterno della base, disintegrandolo. Subito dopo l'esplosione sembra confermato che alcuni terroristi, scesi da un veicolo che seguiva il camion ed intenzionati a penetrare nel *compound* a seguito del forzamento dell'ingresso principale, visto il fallimento del piano di attacco, si sono rifugiati all'interno di una palazzina antistante la base da cui hanno iniziato un fuoco diretto sugli edifici del PRT. La deflagrazione causata dall'esplosivo portato dal camioncino ha provocato rilevanti danni ad una palazzina utilizzata dall'Unità di cooperazione civile e militare nazionale ed il crollo di un'altana. L'esplosione ha causato la morte, oltre che dell'attentatore, anche di un interprete afgano che si trovava all'esterno della base e, unitamente alle conseguenze del crollo delle infrastrutture, è stata causa del ferimento dei nostri militari che non sono risultati colpiti da armi da fuoco. Alle successive ore 8,59 italiane, ovvero alle 11,29 locali, immediatamente dopo l'attacco dinamitardo, ha preso avvio l'attacco a fuoco da parte degli *insurgent* che si erano introdotti negli edifici adiacenti il PRT e, in particolare, in una casa in costruzione, raggiunti dagli altri che sarebbero dovuti entrare nel portone principale. Il fuoco veniva condotto con l'impiego di armi portatili, bombe a mano e razzi anticarro RPG. Un razzo ha colpito il veicolo civile Toyota in uso al comandante del PRT che, prendendo fuoco, ha provocato l'incendio di un ufficio adiacente. Al termine dello scontro e del rastrellamento venivano ritrovati due giubbotti esplosivi che non era stato possibile utilizzare da parte dei terroristi. A seguito dell'esplosione è stato immediatamente attivato il piano di difesa ed il personale ha raggiunto le postazioni predefinite per la reazione. Personale italiano presente nel PRT ha reagito all'attacco con le armi in dotazione ingaggiando gli obiettivi avversari rappresentati dagli *insurgent* localizzati negli edifici vicini al PRT. A seguito dell'evento, il comando del *Regional Command West* ha disposto l'immediato intervento di elicotteri tipo A129 Mangusta per il supporto di fuoco, di altri elicotteri multiruolo per l'evacuazione del personale ferito,

hanno rapidamente cinturato l'area ingaggiando a loro volta le sorgenti di fuoco avversarie. In sintesi, in tempi successivi, sono intervenuti nostri militari in servizio di guardia e della Forza di reazione immediata del PRT, le Forze speciali italiane e statunitensi Inoltre, il personale italiano specializzato ha proceduto alle operazioni di bonifica e messa in sicurezza all'interno del *compound*. All'esterno, personale nazionale e statunitense è intervenuto, unitamente alle Forze di sicurezza afghane nella palazzina da dove proveniva l'azione di fuoco e per la disattivazione di ordigni esplosivi. Infine, il personale delle Forze di polizia e di sicurezza afghane ha provveduto per la messa in sicurezza e la bonifica della zona circostante il PRT. Le attività di rastrellamento si sono concluse alle ore 17,25 locali.

Non è stata confermata invece la notizia di un altro attacco condotto contro la sede del governatore di Herat, che era circolata in un primo momento. A seguito dell'esplosione e del crollo della palazzina CIMIC, si è registrato il ferimento di 5 militari italiani, più uno in stato di *shock*. I feriti sono stati

realizzato il ferimento di quattro civili, di cui uno sloveno e tre afgani. Vi ho già anticipato che nessuno di loro è stato colpito da proiettili, ma tutti da schegge e macerie dovute all'esplosione. In particolare, il ferito più grave è un capitano, che ha riportato una lesione pancreatica post-traumatica, una frattura vertebrale dorsale e una contusione lobo frontale.

inoltre catturato l'attentatore che ha fatto esplodere l'ordigno nei pressi dell'ospedale, pochi minuti prima dell'attacco al *compound*. Al termine dell'evento sono stati contati 5 deceduti e 32 feriti tra i locali afgani, e uno dei feriti è successivamente deceduto. Anche a loro, oltre che alle famiglie dei nostri militari e al popolo afgano, va la nostra vicinanza e la nostra commossa solidarietà. alcune breve considerazioni anche sull'Afghanistan, che in questo momento è interessato da una fase cruciale, quella della transizione delle responsabilità di sicurezza dalle forze ISAF a quelle afgane. Herat rappresenta senza dubbio il simbolo del processo della transizione nella regione Ovest ed appare evidente che l'attentato sia parte di una strategia della tensione rivolta contro tale processo. Proprio nella giornata dell'evento di cui vi sto riferendo, il 30 maggio, era in atto la Conferenza nazionale afgana

D'altra parte, nonostante fosse chiaro che questo evento avrebbe potuto sicuramente portare ad azioni ostili, non possiamo rimproverare nulla perché tutte le misure di sicurezza possibili erano state approntate nella regione Ovest. c'è un'altra zona considerata tranquilla, quella sotto il comando tedesco, che aveva subito proprio nei giorni precedenti un altro attentato in cui era rimasto coinvolto un generale tedesco. Mettendo Mettendo insieme i due eventi, è chiaro che la strategia è quella che ho appena enunciato, ossia tentare di bloccare la fase di transizione che evidentemente è quella che più di ogni altra preoccupa gli *insurgent* afgani, talebani e quant'altro. Sul piano tattico la valutazione dei nostri militari è che l'attacco sia comunque fallito (dal loro punto di vista, dal punto di vista di chi lo ha organizzato e condotto), nonostante i feriti e i morti afgani che ha prodotto. Evidentemente l'obiettivo era assai diverso e va registrato che tutti coloro che hanno condotto l'attacco sono stati neutralizzati. essere segnalato che anche in questo caso chi ha pagato il prezzo più alto sono stati i civili inermi, coinvolti in maniera sconsiderata e irresponsabile dai terroristi in questo attacco, che hanno pagato con la vita. Occorre sottolineare un dato, che è l'unico aspetto positivo di questa ulteriore drammatica vicenda che si aggiunge ai tanti lutti e ai tanti momenti di tensione che abbiamo dovuto commentare anche in quest'Aula. Tutta la dinamica che vi ho illustrato consente di esprimere un giudizio estremamente positivo sulla accresciuta capacità reattiva della polizia e dell'esercito afgano, che sono stati addestrati dai nostri militari e hanno dimostrato anche in tale occasione di aver acquisito la capacità di stare sul terreno e di rispondere alle ostilità, vicina alla professionalità del contingente internazionale. Questo è un titolo di vanto per gli istruttori, ma è soprattutto un motivo di conforto per chi, come noi, aspira a rendere operativa e decisiva la fase di transizione, che, secondo le previsioni, potrebbe concludersi nel 2014, con la riconsegna di tutto il territorio afgano al legittimo Governo di quel Paese. Certamente non è possibile escludere che in futuro si verifichino altri eventi similari; anzi, devo dirvi che la fase è tale per cui ogni ora siamo in contatto, perché temiamo la possibilità di ripetizioni di atti del genere. Ma, dall'altro lato, la capacità di reazione mostrata dalle nostre forze e da quelle afgane costituisce un valido presupposto perché il progetto di trasferire la responsabilità di sicurezza nelle loro mani possa essere completato positivamente. Un altro elemento che bisogna segnalare è che l'attacco non è stato disposto contro un dispositivo militare; si è trattato anzi di un attacco contro un organismo di ricostruzione, che tende ad assicurare condizioni di vita migliori al popolo afgano (ospedali, scuole, acqua, condizioni di socializzazione). Questo dimostra da un lato il lavoro che è stato fatto e, dall'altro, che gli *insurgent*, i terroristi, temono più di ogni cosa la nostra capacità di conquistare il cuore e le menti dei cittadini afgani. Non si spiega altrimenti la volontà di attaccare non una base militare, ma un luogo nel quale i cittadini hanno solo dato amicizia, solidarietà, vicinanza, con forte aiuto. Per concludere, credo che quello dei giorni scorsi sia stato evidentemente un disperato tentativo degli *insurgent* di impedire questo processo, che è in atto, che noi consideriamo avanzato in Afghanistan e che ci consente di sperare bene per il futuro, di cui però non vi nascondo i pericoli. Essi non diminuiranno; anzi, con l'avvicinarsi dell'obiettivo è prevedibile che

A loro, a questi ragazzi, alle ragazze, ai loro comandanti, che così bene stanno cercando di condurre avanti questa difficilissima missione, vanno la mia e - sono convinto - anche la vostra vicinanza e la vostra solidarietà.

Anche il Partito Democratico naturalmente si associa alla solidarietà che il sottosegretario Crosetto ha appena espresso ai soldati che sono rimasti vittime di questi attentati e alle alle loro famiglie. Desideriamo esprimere allo stesso tempo una forte preoccupazione, perché riteniamo che le modalità con le quali questi attentati sono stati perpetrati segnalino la volontà di alzare il livello dello scontro. Ci preoccupa particolarmente l'attentato

rappresenta il tramite attraverso il quale creare un'unificazione tra il mondo militare (e quindi le varie articolazioni dei Paesi presenti) e la società civile.

di informale non c'è niente - l'eventualità di una riduzione della presenza dei nostri militari sia in Afghanistan che in Libano.

ha esortato - non credo che questo verbo costituisca una forzatura - i Paesi che compongono l'UNIFIL a non abbassare la guardia. guardia. Noi, che naturalmente non siamo guerrafondai e che rispetto alla necessità di essere presenti nei teatri internazionali ci poniamo davvero con lo spirito di portare avanti missioni di pace e non di guerra, riteniamo però che non ci possa e non ci debba essere leggerezza nel trattare queste materie. In particolare, riteniamo che non sia consentito che la leggerezza venga espressa magari dallo stesso Presidente del Consiglio, il quale, a seconda dei rapporti che intercorrono tra lui ed il capo riconosciuto della Lega, declina le proprie posizioni più per sedare eventuali risse che non per fare

decreto sulle missioni internazionali senza che il Parlamento sia stato preventivamente coinvolto. Le chiediamo pertanto di farsi portavoce nei confronti del signor Ministro, affinché almeno questa volta,

I due attentati che si sono susseguiti così a breve distanza l'uno dall'altro, prima in Libano e poi in Afghanistan, sembrano avere la stessa radice. Infatti, è sempre più forte il sospetto che dietro a questi attacchi vi sia un chiaro messaggio dissuasivo nei confronti delle nostre truppe a stabilire un contatto diretto con le popolazioni locali. *(Brusìo).* Signor Presidente,

In Libano sei militari italiani della missione UNIFIL sono rimasti feriti in seguito a un attacco contro i mezzi dell'ONU. più accreditata è che dietro all'attentato ci possa essere un messaggio rivolto alla comunità internazionale, impegnata proprio a condannare la dura repressione siriana. I soldati italiani sono in Libano dal settembre 2006 nell'ambito della missione Leonte, che fa parte dell'intervento ONU denominato UNIFIL. L'Italia partecipa alla missione internazionale con un contingente di 1.780 militari. Appena tre giorni dopo l'attentato in Libano quattro aggressori hanno sferrato un attacco nei pressi del Centro per la Ricostruzione Provinciale di Herat, unità NATO nell'Afghanistan occidentale, gestita da soldati e da civili italiani. Secondo le *intelligence* italiane e americane, anche questo assalto, che ha lasciato feriti cinque militari italiani, sarebbe servito per spezzare il legame tra i militari in azione di pace e il popolo civile. Il timore che aleggia ora è quello che altri possibili attentati contro obiettivi dell'esercito di pace siano già pianificati, anche in virtù del fatto che da circa un mese sono in forte aumento alcune piccole operazioni di intimidazione e continue sparatorie. *(Brusìo).* Signora Presidente, mi scusi, consegno l'intervento.

Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, innanzitutto intendo esprimere ancora una volta, una volta, personalmente e a nome del Gruppo dell'Italia dei Valori, solidarietà alle famiglie di tutte le vittime degli ultimi attacchi avvenuti in Afghanistan e in Libano. Desidero altresì ribadire la vicinanza e la gratitudine alle Forze armate, impegnate ogni giorno con dedizione, passione e impegno nelle missioni internazionali Mi dispiace dover rilevare - e non lo faccio con polemica, ma solo perché credo che sia necessario - che come sempre il Governo e i relativi rappresentanti di turno si occupino dei nostri ragazzi impegnati in queste difficili missioni quasi esclusivamente in occasione di attentati e attacchi, o comunque di eventi caratterizzati da una certa gravità. La ringrazio quindi, signor Sottosegretario, per le informazioni che ha voluto fornire circa la ricostruzione degli eventi che nell'arco di pochi giorni hanno interessato i nostri militari. Credo però che, a prescindere dagli ultimi gravi incidenti, il Governo, in entrambe queste situazioni, non abbia presentato al Parlamento una posizione politica chiara e seria, soprattutto a fronte dei forti cambiamenti che stanno avvenendo in quei Paesi. Ricordo in proposito che è dall'inizio della legislatura che si discute di una legge quadro sulle missioni internazionali. Ve ne sono diverse, depositate in entrambi i rami del Parlamento (una peraltro presentata dallo stesso Governo), ma ancora procediamo a rinnovare con decreti legge la nostra partecipazione a queste missioni, continuando purtroppo a non avere un programma! È evidente come stiano aumentando i pericoli per i nostri soldati e per le nostre truppe e come gli ultimi gravi attentati avvenuti contro le nostre Forze armate, sia in Libano che in Afghanistan, pongano con urgenza la necessità di una riflessione sul ruolo svolto dai nostri militari in quelle regioni. Dico questo non solo perché siamo preoccupati per l'incolumità dei nostri ragazzi, ma anche perché siamo convinti che la presenza delle nostre Forze armate in scenari di guerra o, comunque, in aree estremamente conflittuali, debba essere una presenza sempre ragionata, responsabile e attenta ad ogni cambiamento, non certo con l'attenzione che i colleghi stanno ponendo a questo dibattito. L'Italia, di fronte a questa situazione, risulta essere poco presente e attenta nonostante, tra l'altro, il nostro contingente in Libano sia ancora oggi il più numeroso. Per quanto riguarda l'Afghanistan, la posizione dell'Italia dei Valori è da sempre stata chiara. Abbiamo ribadito più e più volte il nostro convinto no alla permanenza delle truppe in Afghanistan. Lo abbiamo fatto dall'inizio della legislatura chiedendo una *exit strategy*, ovviamente negata e poi considerata la soluzione migliore addirittura dal presidente Obama e dalla NATO.

una percezione chiara della grave realtà di quel Paese e che ogni giorno il rischio per i nostri militari si fa sempre più elevato. È ora di prendere delle decisioni serie e responsabili nei confronti non solo di tutti i militari impegnati nelle missioni, ma anche nei confronti di tutto il Paese. È necessario, conseguentemente, rivalutare con attenzione e serietà la partecipazione del nostro contingente in queste missioni internazionali.

in Afghanistan ogni minaccia è un fantasma che ti segue e ti perseguita dappertutto. Vorrei chiedere al Governo

Signora Presidente, signor Sottosegretario, negli ultimi dieci giorni in alcune delle zone dove sono impegnati i nostri militari si sono succeduti tre attentati, come è stato ricordato. Il primo il 27 maggio

Gli attacchi contro i nostri militari lasciano sempre tutti sgomenti. Anche noi vogliamo esprimere la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime e ai feriti, augurando loro una pronta guarigione. Gli attentati subiti in questi anni, che purtroppo negli ultimi mesi si sono intensificati proprio quando la transizione, soprattutto in Afghanistan, appare più vicina, ci rafforzano nella convinzione che la presenza militare italiana non è stata inutile, ma anzi è stata utile e proficua. Tuttavia, a nostro giudizio, si pone con forza la questione di un riequilibrio progressivo della presenza italiana nei teatri di intervento, che ad oggi non sono più considerati strategici. Non vogliamo dire niente di nuovo dal momento che una riflessione in questa direzione è stata compiuta nei giorni scorsi anche dai ministri Frattini e Calderoli. A nostro avviso, però, è arrivato il momento di dare un segnale politico che non può e non deve essere interpretato come una defezione: i militari impegnati nelle missioni all'estero hanno e continueranno ad avere tutto il nostro sostegno. Ci sembra, però, che un riequilibrio delle presenze dei nostri militari nei vari scenari appaia oggi una decisione di maturità e di responsabilità. di responsabilità. Si potrebbe seguire l'esempio, soprattutto per il Libano, del modello che è già stato attuato con le missioni nei Balcani: ad un progressivo consolidamento pacifico della situazione si è proceduto con un graduale riequilibrio delle forze in campo. Dal momento che lo stesso ministro La Russa ha evidenziato che in futuro, soprattutto in Afghanistan, i rischi per i nostri militari non diminuiranno, auspichiamo che lo stesso processo di transizione venga accelerato e monitorato con maggiore attenzione rispetto ad oggi. Certo, sappiamo bene che l'Italia è parte di una coalizione e che le decisioni vanno contemperate nel quadro di un'alleanza, ma è ora che il Governo e la nostra diplomazia contribuiscano ad un salto di qualità. È evidente ed apprezzabile che un negoziato politico-diplomatico in tutta la regione venga messo in atto al più presto possibile; un negoziato che però deve proseguire e procedere di pari passo con una presenza militare riequilibrata nelle sue dimensioni per ottimizzare il nostro ruolo e per far sì che non ci si debba ritrovare così spesso con il Governo a relazionare su attentati e con le forze parlamentari ed i politici ad esprimere costernazione e solidarietà per le vittime.

Credo che dobbiamo scandire una tempistica assieme alla NATO e mettere in condizione il presidente Karzai e il Governo afgano

- dall'ultima sessione dell'Assemblea primaverile della NATO, dove ho rilevato che è cominciato a passare in alcuni Paesi il concetto che,

*(PdL)*. Signora Presidente, onorevoli Sottosegretari, onorevoli colleghi, desidero ringraziare il sottosegretario Crosetto

coinvolte. Quando i nostri militari impegnati in missioni umanitarie all'estero rimangono vittime di attentati, all'inizio veniamo colti da sentimenti di angoscia e di impotenza, mentre attendiamo notizie rassicuranti sul numero e sulle condizioni dei militari coinvolti; immediatamente ci immedesimiamo nella condizione delle loro famiglie, che vivono quotidianamente l'angoscia che i loro congiunti possano subire lesioni o perdere la vita nell'esercizio del dovere.

In un secondo tempo questi sentimenti sfociano inevitabilmente nel desiderio di far tornare a casa tutti i nostri militari, ponendo fine a missioni che diventano di giorno in giorno più insidiose, cosicché si susseguono invocazioni al ritiro delle truppe o perlomeno ad una riduzione cospicua o per nulla graduale dei contingenti dislocati. E queste invocazioni tentano tanto più noi parlamentari che sentiamo il peso delle decisioni assunte, allorché siamo chiamati a deliberare l'invio delle truppe all'estero nei teatri più caldi del pianeta. Noi riteniamo che un ritiro, come correttamente evidenziato dal ministro La Russa e ribadito dal sottosegretario Crosetto, possa avvenire in termini graduali ma con grande prudenza, perché questi scenari internazionali non hanno ancora guadagnato la capacità di una democrazia interna, alla quale noi siamo

Dal 27 maggio abbiamo invece scoperto di essere vulnerabili anche nel vicino Libano ed abbiamo accarezzato l'idea di ridurre o di azzerare anzitempo anche lì il nostro impegno. impegno. Vorrei cogliere l'opportunità di questo intervento per ribadire con forza a nome del Gruppo che mi onoro di rappresentare che in questi momenti non possiamo chiedere o desiderare un disimpegno dell'Italia dal Libano o dall'Afghanistan o da qualunque altro Paese ci veda impegnati, e questo perché la politica e la difesa della democrazia, ahimè, in un mondo globalizzato,

È chiaro che una riduzione del nostro impegno può e deve avvenire solo a seguito dell'accertata cessazione delle ragioni che lo hanno determinato, e che sono essenzialmente di natura umanitaria e di ripristino dei valori democratici più basilari. E non mi sembra proprio che ciò possa dirsi in un momento in cui quasi tutti i Paesi mediorientali sono connotati da una forte instabilità e i tentativi, più o meno coraggiosi, della popolazione di emanciparsi

mai come in quella che viene definita, forse in maniera un po' frettolosa ed ottimistica, la primavera araba bisogna essenzialmente assicurare nel Medio Oriente e nel lontano Oriente la continuità dell'impegno della comunità internazionale, in seno alla quale il ruolo di tutto rispetto che l'Italia è riuscita a ritagliarsi si deve soprattutto al lavoro svolto dalle nostre Forze armate dai loro vertici, universalmente apprezzati per la professionalità, generosità e umanità con cui svolgono i propri compiti. A loro va la nostra ammirazione ed il nostro sentito ringraziamento.

Nella seduta antimeridiana di oggi, dopo avere esaminato l'articolo 1 e gli emendamenti ad esso riferiti, l'Assemblea ha convenuto, su richiesta del rappresentante del Governo, di sospendere brevemente l'esame del disegno di legge.

il Governo ha esaminato anche tecnicamente il testo degli articoli del disegno di legge che rimanevano da approvare e le conseguenze della mancata approvazione dell'articolo 1, così come proposto

esattamente come era già successo con i tre articoli usciti da questo testo ed entrati in altri provvedimenti, la gran parte delle misure che dobbiamo discutere ed approvare in quest'Aula ha una valenza in sé, a prescindere dall'articolo 1. Certamente - non intendiamo negarlo in nessun modo, anche perché l'abbiamo detto immediatamente e con grande lealtà nel momento in cui è stato bocciato l'articolo 1 - rimane il problema che quell'articolo inseriva, finalizzava e contestualizzava tutto il resto dell'articolato nell'ambizione, che tutti noi abbiamo, di dare un coordinamento a tutte queste materie.

Voglio dire con grande franchezza che noi avremmo potuto meditare più a lungo la stesura di questo emendamento,

la corruzione - andasse rafforzata l'autorevolezza e la qualità della struttura di coordinamento, rendendola di fatto più rispondente alle aspettative emerse dalla discussione in Aula. l'emendamento prevede la costituzione di un comitato che, una volta insediato, si avvarrà delle strutture del Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; composto dal procuratore generale della Corte di cassazione, dal presidente del Consiglio di Stato, dal procuratore generale della Corte dei conti, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal capo della Polizia, dal comandante della Guardia di finanza, dal presidente dell'Autorità nazionale di vigilanza sui lavori pubblici, e via via da tutta una serie di soggetti che hanno ruoli di alta dirigenza o di responsabilità diretta proprio nell'attuazione delle politiche di contrasto alla lotta alla corruzione ed anche anche delle politiche di prevenzione e repressione di tutti quei fenomeni che possono favorire, anche in termini ambientali, eventi che determinano conseguenze molto gravi, tra cui anche la corruzione.

Di conseguenza, spetterebbe a questo comitato elaborare a livello nazionale e internazionale l'attuazione dei principi di cui all'articolo 5 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e tutto quello che ne consegue. [**Presidenza del presidente

ore. Innanzitutto, non dobbiamo dimenticare che questa formulazione dovrebbe essere piuttosto rassicurante rispetto all'idea che personalità del genere, riunite in un comitato, possano subire una qualsivoglia forma di condizionamento. È evidente che, se così fosse, non potrebbero permanere nemmeno negli incarichi che ricoprono attualmente. Tanto per essere chiari, dubito che si possa considerare sottoposto a qualche forma di influenza il Comandante dell'Arma dei carabinieri o il Presidente della Corte dei conti. Ciò sarebbe abbastanza inverosimile da sostenere, oltre che offensivo nei loro confronti.

alle stesse aspettative che abbiamo suscitato. Quindi, da questo punto di vista, mi auguro che si colga anche in tale emendamento lo sforzo del Governo di arrivare a detto risultato. Il Presidente del Senato ha voluto con grande forza che ci trovassimo in quest'Aula

che ringrazio per il garbo, ma non per il merito. Quest'Aula ha fatto due votazioni questa mattina: con il primo voto è stato bocciato l'emendamento del senatore Malan; con il secondo è stato bocciato l'articolo 1 del disegno di legge. ciò che è stato bocciato è il sistema con il quale viene radicata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Autorità - o chiamatela come volete - che deve governare il controllo Questo è il punto. E, se questo è il punto, non è ammissibile né proponibile alcun emendamento che riproduca questo sistema. Al sottosegretario Augello, che per inciso, e con grande abilità retorica, dice che non è possibile ricorrere al sistema dell'Autorità indipendente (come l'articolo 6 della Convenzione ONU sulla corruzione del 2003 impone), del 2003 impone), io chiedo quali siano - ohibò! - le ragioni di questa impossibilità, che peraltro, come possibilità positiva, viene invece prevista in altri disegni di legge presentati e abbinati a questo provvedimento. Mi resta oscuro perchè noi dobbiamo o dovremmo contravvenire, o proponiate di contravvenire all'articolo 6 della Convenzione ONU, per creare un carrozzone - mi perdonino le insigni personalità che verrebbero a comporre questo organismo - che resta saldamente E voglio ancora aggiungere che non solo abbiamo dalla nostra l'articolo 97, secondo comma, del Regolamento del Senato della Repubblica, che appunto dichiara inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato sull'argomento sull'argomento nel corso della discussione, ma abbiamo dalla nostra anche un'altra proposta positiva.

dalle opposizioni e abbinati a questo provvedimento: sono tutti disegni di legge rispetto ai quali io non esprimo nessuna preferenza. Il Governo ritiri il proprio provvedimento, si vada in Commissione, si scelga uno di questi testi come testo base, su questo si costruisca un provvedimento assai più compiuto, profondo, efficace e rispondente alle prescrizioni internazionali Questo è quello che abbiamo voluto dal primo momento, presentando i disegni di legge anticorruzione (ben tre sono quelli del mio Gruppo), sollecitando in ogni sede e con ogni forma - compresa una lettera diretta a lei, presidente Schifani - la discussione del provvedimento anticorruzione, presentando noi il disegno di legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo ed impegnandoci in ogni modo perché l'Italia abbia una disciplina anticorruzione che faccia onore alla necessità di liberare il nostro sistema dalla corruzione. Siamo pienamente consapevoli dei guasti, non misurabili solo con il metro del codice penale, che la presenza della corruzione reca al nostro sistema, alle competitività del Paese, alla libertà dei nostri mercati e alla possibilità delle nostre imprese di muoversi secondo regole chiare e definite. Perché volete ostinarvi? Il vostro disegno di legge è sbagliato, ed è stato bocciato per due volte dall'Assemblea del Senato. L'opposizione, il più grande partito dell'opposizione, stende davanti voi il tappeto rosso della possibilità di avere, in tempi brevi, una disciplina efficace e rispettosa

noi saremo costretti ad esperire ogni mezzo perché si eviti che questo Senato torni a discutere di un argomento che ha già bocciato.

su questo tema, ad assumere insieme a voi, portandone la responsabilità? Purché queste siano chiare, serie, efficaci e rispettose della legalità internazionale.

che sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato sull'argomento nel corso della discussione. stabilisce che il Presidente del Senato, nell'interesse della discussione, può decidere l'accantonamento e il rinvio alla competente Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti, stabilendo la data nella quale la discussione degli stessi dovrà essere ripresa in Assemblea. Il testo che il Governo con questo emendamento intende sottoporre all'Aula è oggettivamente inammissibile, ai sensi delle disposizioni che ho citato, per una serie di ragioni, signor Presidente. La prima riguarda il merito ed il contenuto: l'Aula ha deciso che non è possibile che l'Autorità anticorruzione sia gestita dall'Esecutivo e dalla Presidenza del Consiglio, ma che debba essere un'autorità terza. luogo, l'Aula ha deciso che quest'Autorità terza deve avere una serie di poteri coercitivi, penetranti rispetto al tessuto dell'amministrazione su cui si ritiene vi siano rischi di corruttela. terzo luogo, l'Autorità devo essere indipendente e non deve interferire con altri poteri dello Stato, per cui l'idea che il Governo ha preannunziato nel suo emendamento di mettere dentro il procuratore generale della Corte di Cassazione, la Corte dei conti, i Carabinieri a cavallo, la Guarda di finanza e la Guardia forestale, evidenzia evidenzia profili di incostituzionalità del testo, perché la funzione della norma ed il contenuto della Convenzione ONU dicono esattamente il contrario. *(Applausi dai

lei deve assumersi una responsabilità, perché lo prevede il Regolamento, non solo con riguardo all'evidente ed oggettiva inammissibilità della proposta del Governo, ma anche con riferimento alla circostanza che, poiché l'articolo 1 è l'articolo principe, quello cioè che dà attuazione alla Convenzione ONU, senza di quello non possiamo andare avanti. Lei

ho compreso la comunicazione del Sottosegretario, ma da profano dei lavori d'Aula, avendo un'esperienza limitata, sono a chiedermi cos'è l'emendamento. In base alle scarse letture che ho potuto fare, l'emendamento è qualcosa che si inserisce per

di legge che parlano di questo argomento, ma qui stiamo discutendo un testo di legge che parla di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Mi sembra un argomento un po' diverso, mentre ci sono

si è lavorato puntando naturalmente ad assumere come testo base il disegno di legge del Governo, ma nel momento in cui la Commissione non ha esaurito il suo lavoro, si è arrivati in Aula con sei disegni di legge, non con uno solo. All'ordine del giorno sono sei disegni di legge. Poi è ovvio che, essendo la materia connessa, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, si procede con un esame unitario,

noi non potremo più ripetere perché è troppo nuova. Abbiamo sbagliato noi a insistere per la calenderizzazione? Ha sbagliato la Commissione bilancio a impiegarci sette mesi per darci i pareri? Si è creata

però facciamolo bene. Ci sono le condizioni per farlo bene, anche alla luce di quello

Signor Presidente, gli interventi del senatore Li Gotti sono sempre interessanti, anche se francamente questa volta ha parlato per un quarto d'ora, ma si è capito poco. Si è voluto usare più il politichese che

come invece si sono svolte oggi le cose in quest'Aula, mi sembra evidente che le opposizioni abbiano voluto arrivare a questa calendarizzazione urgente, tant'è che siamo arrivati in Aula senza i relatori e dunque senza che fosse terminato l'esame del provvedimento in Commissione, perché

opposizioni)*. Si può discutere di tutto, ma lo si deve fare in maniera costruttiva e senza prendere in giro, alla fine, gli elettori e i cittadini che stanno seguendo i lavori di quest'Aula attraverso le trasmissioni radiofoniche e televisive.

credo che affermare che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, il Presidente del Consiglio di Stato,

pensiamo invece che, come al solito, le opposizioni dicono una cosa, ma in Aula fanno esattamente il contrario. Il loro scopo è solo quello di avvelenare il clima politico e non invece di arrivare all'approvazione di un provvedimento che l'intero Paese aspetta da tempo.

dei normali rapporti tra l'Aula e il Governo. Insomma, si può anche provare a fare qualche forzatura, ma qui siamo ad un voto d'Aula che, dopo qualche ora, viene in sostanza completamente capovolto con la presentazione di un articolo aggiuntivo. Tuttavia, il provvedimento ha un suo significato, una sua importanza per il Paese.

questa parte del provvedimento e domani mattina tornare in Aula. È chiaro che ci vuole uno sforzo per venire incontro alle esigenze di contenuti che l'Aula ha

di strumenti contro la corruzione. Ciascuno quindi presenterà emendamenti, anche il Governo naturalmente, che tiene a quelle misure recate dagli altri articoli del suo disegno di legge, sulla cui validità, come dire, io mi voglio esprimere, perché ci sono anche suggerimenti positivi. Diamo pertanto un termine ai lavori della Commissione, così rispettiamo tutti il nostro impegno, e approfittiamo del per discutere subito il provvedimento che ratifica la Convenzione di Strasburgo in materia di corruzione, esitato ieri dalle Commissioni riunite 2a Daremo così - mi pare - la massima prova della volontà del Parlamento italiano di occuparsi di questo tema, non commetteremo smarginature, non ridurremo una cosa così complessa a una dichiarazione di ammissibilità o di inammissibilità, scaricando - mi si consenta il termine - sul Presidente del Senato la sorte di questa questione e ciascuno di noi potrà così trovare il modo di contribuire ad una legislazione seria ed efficace.

Signor Presidente, anche cogliendo la sostanza dell'intervento della presidente Finocchiaro, a me pare che la situazione sia la

C'è una proposta venuta da senatori D'Alia e Bruno di investire la Commissione di questo approfondimento e di cogliere gli elementi di compatibilità o meno del nuovo testo non solo con il testo base, che rimane come testo di riferimento, ma anche rispetto agli aspetti formali che sono stati richiamati. Un passaggio in Commissione limitato a questo aspetto consentirebbe due cose: innanzitutto, non metterebbe l'Aula di fronte alla necessità di prospettare un braccio di ferro regolamentare;

soprattutto da parte delle forze dell'opposizione. A me sembra che questi siano una proposta e un margine offerti dal dibattito che possono essere utilmente colti dalla maggioranza, ma anche da settori dell'opposizione. Tale portarci ad una soluzione compatibile con le esigenze di urgenza che sono state prospettate, più da voi che da noi, e anche con le legittime esigenze di approfondire la compatibilità e la effettiva novità

È stata sempre intenzione di questa Presidenza fare in modo di essere sensibile alle richieste sia di maggioranza che di opposizione tutte le volte in cui queste istanze erano finalizzate a un dibattito su temi sensibili del Paese.

Questo disegno di legge è stato presentato dal Governo un anno e due mesi fa; è stato in effetti fermo per alcuni mesi in Commissione perché mancavano dei pareri della Commissione bilancio. Vi sono state delle sollecitazioni...

Su parecchie sollecitazioni dei Gruppi di opposizione, che recentemente non hanno più votato il calendario,

Ma è chiaro che questo aspetto sconta in Aula un deficit di procedibilità e di organicità di lavoro (non dobbiamo nascondercelo), perché anticorruzione che giunge in Aula senza un relatore, con un testo base soltanto, con una relazione del Presidente della Commissione sicuramente non consente, non tanto alla Presidenza, bensì a chi deve partecipare al dibattito e votare, una visibilità organica ed ampia

con un'articolazione accettabile e che tocchi i vari gangli, per esempio, nella fattispecie, della corruzione, la sua disciplina e l'istituzione di organismi finalizzati al contrasto alla corruzione in un ambito più ampio di articolazione.

che sia possibilmente la più condivisa. Il mio sforzo, e credo lo sforzo di tutti noi, è, quanto meno su temi come l'anticorruzione, di instaurare un clima d'Aula e una responsabilità collegiale che porti a scontrarci e a confliggere sui contenuti, ma non sul procedimento, e principalmente non sulla compiutezza di un disegno di legge. Preferirei evitare che si possa dire che dal Senato è uscito un testo anticorruzione monco. Sarebbe questa una sconfitta di tutti. Non sta a me entrare nel merito se sia monco o meno senza l'articolo 1, però voglio esperire questo tentativo convocando la Conferenza dei Capigruppo per le ore 18. Spero che da essa possa scaturire una decisione unanime sull'andamento dei lavori, nell'interesse della trattazione al meglio di un tema sensibile come la lotta alla corruzione, tema che sta a cuore di tutti gli italiani e certamente di tutti i senatori che compongono quest'Assemblea.

in Conferenza dei Capigruppo è stato affrontato il delicato tema della rivisitazione di quello che era l'argomento affrontato in un certo modo, con una certa ottica, dall'articolo 1 oggi bocciato dall'Aula, cioè quello della modalità di un'azione di controllo sul contrasto alla corruzione, nell'ambito della pubblica amministrazione e non. Ci si è sforzati tutti, con grande senso di responsabilità, di dare innanzitutto un segnale al Paese, ossia che su temi sensibili il Parlamento non si tira indietro e va avanti lavorando, facendo in modo che, se vi sono dei temi che meritano un approfondimento e possibilmente una condivisione di posizioni tra le parti, questi argomenti possano essere stralciati, seppur per poche ore, per poter essere riesaminati in un'Aula che lavora secondo tematiche e scelte condivise. Da qui è nata la scelta e l'intesa secondo la quale domattina il Governo, ad inizio dei lavori, presenterà un emendamento che, riprendendo il tema trattato all'articolo 1, faccia proprie le osservazioni di fondo dell'opposizione in ordine alla configurazione di un organismo autonomo e indipendente cui devolvere la responsabilità del controllo sull'attuazione delle norme anticorruzione e sull'andamento della corruzione nella pubblica amministrazione e dei singoli comportamenti dei singoli soggetti. Questo chiedeva l'opposizione, cioè l'istituzione di un'ulteriore figura rispetto alla proposta del Governo. Vi è stata un'accettazione di questa richiesta ad opera dei rappresentanti del Governo che hanno partecipato alla Conferenza dei Capigruppo e, attraverso questa mia iniziativa e quest'opera di mediazione, posso confermarvi due cose: che quest'Assemblea domattina continuerà ad occuparsi del disegno di legge anticorruzione, così come la prossima settimana (adesso vi darò lettura del nuovo calendario); che domattina questo Presidente, una volta acquisito il nuovo emendamento del Governo, lo trasmetterà alle competenti Commissioni Commissioni perché lo possano discutere e possano arrivare ad un voto unanime. Questa è l'intesa che già nasce dal contenuto dell'emendamento, che introduce una nuova figura richiesta dalle opposizioni; quindi, lo deferirò immediatamente alle Commissioni competenti perché queste possano esitarlo e rimandarlo in Aula la prossima settimana.

Io non posso che compiacermi di questo esito, perché è una tangibile dimostrazione che, quando vi è un po' di buona volontà da parte di tutti, grande senso di responsabilità, come abbiamo dimostrato, a volte riusciamo a dimenticare (non il sottoscritto: maggioranza, opposizione e Governo riescono a dimenticare) quelle conflittualità, quei toni accesi ai quali mi riferisco spesso, lamentandomene, nei miei pubblici interventi ed a far prevalere l'interesse dei cittadini, dimenticando opposizioni preconcette. Di questo sono molto soddisfatto. Ringrazio l'opposizione, il Governo e la maggioranza, perché credo che, al di là delle posizioni diverse nel merito del contenuto, riusciremo a dimostrare che il Parlamento sa fare la sua parte quando si tratta di affrontare temi delicati come quello della corruzione, che deve essere in cima agli imperativi categorici di ogni buon politico.

al di fuori dei lavori dell'Aula (soltanto questo emendamento e quindi, senatore Berselli e senatore Vizzini, soltanto questo tema), dove si